la tutela dell'ordine pubblico, nel quadro di piena collaborazione con il Dicastero competente, quindi il Ministero dell'interno. A tal fine, è stato previsto un cospicuo impiego di personale delle Forze armate. È inoltre noto a tutti che tale attività ha portato a risultati di notevole rilievo incontrando, in particolare, il pieno apprezzamento della popolazione. Con riferimento alla situazione rappresentata dal senatore interrogante, evidenzio che il piano d'impiego del contingente di 3.000 appartenenti alle Forze armate (adottato ai sensi dell'articolo 7*-bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008) ha previsto, per un periodo compreso dal 4 agosto 2008 al 3 febbraio 2009, 2.000 uomini per attività di vigilanza e 1.000 per servizi di perlustrazione e di pattugliamento. Alla luce di questa prima ripartizione, il numero di appartenenti alle Forze armate reso disponibile nella provincia di Napoli

II contingente di 3.000 unità è stato poi integrato con ulteriori 500 militari fino alla data del 31 dicembre 2008 (ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 92 del 2008) al fine di affrontare situazioni di emergenza criminale. Tale aliquota è stata completamente assegnata, a decorrere dal 4 ottobre 2008, alla provincia di Caserta ed utilizzata per compiti di vigilanza fissa a siti e ad obiettivi sensibili, compresi gli assi viari. Successivamente, tenuto conto anche delle sopravvenute esigenze di mantenimento dell'ordine pubblico presso l'isola di Lampedusa, il Capo della Polizia, autorità competente, con decreto del 30 dicembre 2008, ha disposto, a decorrere dal successivo 1° gennaio, l'assegnazione alla provincia di Caserta di un contingente pari a 300 militari (tratti da quelli originariamente assegnati ad altre città), dei quali 115 per esigenze di vigilanza agli obiettivi sensibili e 185 per servizi di perlustrazione e di pattugliamento. ulteriori modifiche al piano d'impiego delle 3.000 unità sono state disposte con decreto interministeriale del 3 febbraio 2009 che ha stabilito un incremento di 55 militari per la provincia di Milano: queste unità sono state recuperate da aliquote precedentemente assegnate a Bari (10 militari), a Roma (10 militari), a Caserta (5 militari) e a Napoli (30 militari). Pertanto, a luglio ultimo scorso, le province di Caserta e di Napoli potevano contare, rispettivamente, su un numero complessivo di 295 e di 154 militari. A Napoli in effetti sono state aggiunte ulteriori 5 unità. Per completezza d'informazione, aggiungo che il Capo della Polizia, con decreto del 30 marzo ultimo scorso, ha previsto l'incremento di 50 militari - tratti dall'aliquota impiegata a Siracusa - al contingente già assegnato (40 unità) per la vigilanza al centro per immigrati di Cagliari. L'attività di controllo straordinario del territorio, attuata con il concorso dei militari, ha consentito di effettuare una capillare vigilanza delle aree maggiormente a rischio, con risultati sicuramente positivi. In considerazione di ciò, l'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ha autorizzato la proroga - per ulteriori due semestri decorrenti dal 4 agosto 2009 - del piano d'impiego di 3.000 militari, con un incremento di ulteriori 1.250 unità, per un totale di 4.250 militari. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 3 agosto 2009 è stato attuato, a decorrere dal 4 agosto 2009, il relativo piano di impiego dei citati 4.250 militari, di cui 2.783 impiegati in attività di vigilanza dei siti e degli obiettivi sensibili e 1.467 impiegati in attività di perlustrazione e di pattugliamento. In particolare, per la provincia di Caserta, è stato previsto un incremento di 30 militari all'aliquota per compiti di vigilanza, configurando un contingente, allo stato, composto da 325 unità, di cui 145 unità per la vigilanza agli obiettivi sensibili e 180 per l'attività di perlustrazione e di pattugliamento. Con decreto del 9 ottobre scorso - avente decorrenza 12 ottobre 2009 è stata altresì disposta la rimodulazione del piano d'impiego dei militari limitatamente ad un incremento di 50 unità, a disposizione del prefetto di Napoli, per l'impiego nei servizi di vigilanza a siti e ad obiettivi sensibili, attraverso la contestuale riduzione di personale militare dai contingenti impiegati presso i centri per immigrati di Bari, Cagliari, Foggia e Trapani.

di realizzare risparmi, dall'altro determina una contrazione significativa del concorso di detto personale nei servizi di vigilanza e di controllo del territorio»,

la ragione per cui, se i risultati sono stati positivi (e nei rapporti delle due prefetture viene evidenziato il contributo dato dalle Forze armate) armate) in questi due territori particolarmente esposti all'aggressione della criminalità - mi riferisco in modo particolare al territorio della provincia di Caserta, dove,

sociali*. Signor Presidente, passo ad illustrare, sulla base dei dati forniti dai competenti uffici dell'amministrazione che rappresento, dall'INAIL e dall'ISPESL, l'atto ispettivo, inerente la materia della sicurezza nel particolare ambito del settore agricolo, agricolo, presentato dalla senatrice Spadoni Urbani. Preliminarmente mi sembra opportuno precisare, al fine di meglio chiarire la ripartizione delle competenze in materia di ispezioni sul lavoro che, ai sensi della vigente normativa (articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni), la vigilanza in materia di salute e sicurezza è demandata, in via generale, alle aziende sanitarie locali e per specifici settori quali, a titolo esemplificativo, quello edilizio o di genio civile, attività comportanti rischi particolarmente elevati, alle Direzioni provinciali del lavoro nonché, per gli aspetti di competenza, ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco ed all'ARPA. Il Governo, in attuazione della normativa di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico sulla sicurezza), ha emanato il decreto legislativo n. 106 del 2009 (ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 123 del 2007) per completare il processo di riforma delle regole in materia di prevenzione degli infortuni in ogni ambiente di lavoro. nel sottolineare che la normativa in parola trova applicazione anche per il settore agricolo, faccio presente che in tale ambito, dal 2001 al 2008, si è registrato un calo significativo degli infortuni pari al 33,8 per cento, in valore assoluto, e al 24,8 per cento, in rapporto al numero di occupati;

Tali risultati sono essenzialmente dovuti ai maggiori investimenti per la formazione e l'informazione degli operatori nonché agli effetti positivi derivanti dall'innovazione tecnologica. Va, comunque, rilevato che gli infortuni di maggiore gravità scaturiscono dall'utilizzo di macchine agricole e forestali che possono essere suddivise in due gruppi a seconda che siano state immesse sul mercato precedentemente o successivamente al 21 settembre 1996; nel primo caso devono rispondere ai disposti di cui all'allegato V

L'accertamento di un'eventuale difformità rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente comporta l'attivazione, in seno al cosiddetto gruppo macchine, di una procedura amministrativa (alla quale prendono parte l'amministrazione che rappresento, il Ministero dello sviluppo economico, il coordinamento tecnico regionale e l'ISPESL) che può sfociare nell'emanazione di un provvedimento di ritiro dal mercato del macchinario. Tutto ciò premesso, non posso non constatare che la sicurezza nell'utilizzo delle macchine e delle attrezzature agricole non dipende solo dalla circostanza che le medesime siano «sicure» o «a norma», ma risulta altresì strettamente correlata alla professionalità dell'agricoltore sostenuta da una forte e corretta cultura della prevenzione. Per tale ragione, allo scopo di migliorare le conoscenze in materia di salute e sicurezza di chi opera nel settore agricolo, sono state intraprese molteplici azioni. In particolare, nell'ambito del Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro (di cui al è stata individuata la necessità di un Piano nazionale di prevenzione agricoltura e silvicoltura per gli anni 2009-2011, al fine di supportare le attività svolte dai competenti organi di vigilanza. In attuazione di tale piano, Regioni e Province autonome, con la collaborazione di ISPESL e INAIL, hanno avviato una serie di attività formative, organizzative e informative allo scopo di: garantire agli organi vigilanti un'anagrafe aggiornata delle aziende agricole; attivare una campagna di controllo sulla applicazione della normativa di sicurezza; promuovere campagne di rottamazione delle attrezzature di lavoro tecnologicamente obsolete; attivare programmi finalizzati alla riduzione dei rischi più gravi; promuovere la formazione dei lavoratori agricoli e degli operatori delle ASL . Inoltre, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, l'accordo del 20 novembre 2008 include tra i destinatari della campagna di comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in fase di avanzata predisposizione a cura del Ministero del lavoro) i datori di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori ed i lavoratori anche del settore agricolo. Nel predetto accordo, inoltre, è previsto il finanziamento, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di programmi di formazione dedicati ai lavoratori stagionali del settore agricolo. Faccio presente, infine, che, l'ISPESL, in collaborazione con le Regioni, sta attuando un progetto (dal titolo «CCM promozione della salute e sicurezza sulle attività agricole, zootecniche e forestali»), approvato e finanziato dall'amministrazione che rappresento, nell'ambito del quale sono previste attività di formazione ed informazione delle figure professionali che, a vario titolo, intervengono nel processo di prevenzione dei rischi aziendali. Il citato progetto prevede inoltre, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, almeno 10.000 controlli da effettuarsi presso le aziende agricole o forestali, finalizzati alla individuazione di eventuali difformità di talune categorie di macchine (fra le quali rientrano quelle oggetto del presente atto ispettivo) ai prescritti requisiti di sicurezza.

vivaddio, sta molto migliorando, dal momento che in questi ultimi anni da 2.000 incidenti siamo passati a circa 130 e ciò significa che qualcosa comincia a funzionare. Tutto ciò di cui ci ha parlato, tutte le azioni pensate e previste dovrebbero aiutare a migliorare ancor di più la situazione. Quello che mi auguro è che tali azioni vengano veramente attuate.

potrà conoscere l'orografia del suolo quanto si vuole, ma basta un sasso per far rivoltare queste macchine pericolosissime, perché non sono stabili. Quindi, ci vuole il controllo

agricoltore, utilizza questi mezzi indispensabili o li mette in mano a persone che devono essere capaci di utilizzarli al meglio; altrimenti, tutte le azioni che si porranno

Presidente, l'interrogazione è del giugno 2009, sicché, francamente, più che leggere la risposta che è stata predisposta dagli uffici, credo di poter rendere una comunicazione più puntuale individuando alcuni passaggi che, nel frattempo, anche a ridosso dell'interrogazione stessa, si sono determinati,

Come giustamente viene indicato ed evidenziato nell'atto ispettivo, la scadenza al 30 giugno dell'appalto Sevel con la cooperativa Albasan nel settore della logistica ha

Con decreto direttoriale n. 47.738 del 27 ottobre 2009 è stato infatti autorizzato, per il periodo 1° luglio 2009-30 giugno 2010, il trattamento straordinario e l'integrazione salariale per crisi aziendale in favore di un massimo di 26 unità dipendenti dalla società Albasan impiegate presso lo stabilimento di Atessa.

ordinaria (CIGO) per carenza di commesse e che è stata autorizzata a fruire un trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga fino al 31 gennaio 2010. Nel frattempo, è in fase istruttoria un programma di investimenti per un valore di circa 143 milioni di euro (per l'esattezza, 143.813.000) nell'ambito di un contratto di programma della Sevel finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Atessa che prevede un incremento occupazionale di circa 100 unità.

ispettivo) il CIPE ha stanziato 300 milioni di euro per il finanziamento di interventi agevolativi volti a fronteggiare le situazioni di crisi in alcune aziende, tra le quali anche la FIAT. Il 7 luglio scorso, in attuazione dell'accordo governativo del 17 aprile 2009, è stata inoltre prevista per la Regione Abruzzo l'assegnazione di 55 milioni di euro finalizzati all'utilizzo di ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella Regione medesima.

la situazione di cui all'atto ispettivo e a garantire, anche nel corso del 2010, gli interventi necessari al fine di non interrompere la tutela ed il sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori.

si è registrata la perdita di 2.200 posti di lavoro; 2.200 famiglie non hanno più una certezza né del presente né del futuro. Da qui la necessità di rivolgere al Governo

assegnato risorse che sono state tolte agli altri cittadini italiani, agli altri contribuenti. Pertanto, conoscere l'esatta strategia di un gruppo industriale che sta ricevendo, come è accaduto nei decenni passati, incentivi e sostegni da parte dello Stato e del Governo credo sia quanto meno un atto necessario e dovuto per dare una prospettiva ai lavoratori e agli operai della Sevel. Ho dei dubbi circa l'esatta protezione che si è pensato di assicurare con gli ammortizzatori sociali. Tenga presente, signor Sottosegretario, che dal 1° gennaio di quest'anno

Ho peraltro dei dubbi anche sul fatto che la crisi attuale che sta vivendo l'agglomerato della Val di Sangro sia dovuta soltanto ad una crisi di commesse,

Il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento delle comunicazioni, riscontrando le diverse segnalazioni di interferenze presentate dalla società GPM Communication, editrice dell'emittente radiofonica «Radio Canale 94 stereo», riguardanti l'impianto di Nova Siri, in provincia di Matera, ha dato incarico al competente ispettorato territoriale di Puglia e Basilicata di predisporre le adeguate verifiche per la constatazione dei fatti. ispettorato, dopo aver segnalato alla suddetta società GPM la necessità di specificare le località interessate dal danno ed i livelli di campo elettromagnetico del segnale interferente, invitava l'emittente stessa a provvedere a redigere un rapporto tecnico su tali presunte interferenze. Gli elementi sopra richiamati sono infatti essenziali per la soluzione delle problematiche rappresentate, in quanto le segnalazioni di interferenze formulate in maniera generica, oltre a non essere in linea con le indicazioni stabilite dall'*International Telecommunication Union* - settore Radiocomunicazioni (ITU-R), non consentono di predisporre, in contraddittorio con le emittenti indicate, come presumibili interferenti, le verifiche tecniche necessarie secondo le procedure di rito. L'ispettorato territoriale di Puglia e Basilicata segnala che, nonostante tale invito, alla data alla data odierna non ha ricevuto alcuna risposta. A seguito di successiva richiesta, da parte della Direzione generale competente, il citato ispettorato ha, comunque, nuovamente avviato la procedura di verifica tecnica dell'impianto in argomento, per accertare lo stato interferenziale,

che ha competenza in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi, è a conoscenza del piano industriale in corso relativo alla cessione da parte di ENI di *asset* e titoli minerari. Si ritiene opportuno illustrare, in premessa, le principali ragioni che hanno indotto l'ENI, che oggi è una delle prime 10 compagnie petrolifere del mondo, a procedere all'attuale riorganizzazione delle proprie attività in Italia. Fin dagli anni '50 del secolo scorso, attraverso un'innovativa politica di incremento delle riserve di idrocarburi e di espansione, rivolta principalmente ai Paesi arabi e a quelli in via di sviluppo, le dimensioni aziendali sono cresciute da quelle di azienda di Stato nazionale, votata principalmente allo sviluppo delle riserve di gas naturale della pianura Padana, a quelle attuali di multinazionale. Nel corso degli ultimi vent'anni sono profondamente cambiati sia lo scenario geo-politico mondiale che le regole europee e nazionali in materia di concorrenza e mercato. La progressiva apertura dei mercati interni dei Paesi dell'Unione europea ha comportato l'abrogazione delle zone di esclusiva nazionali e la progressiva riduzione degli ex monopoli, in contrasto con le regole di libero mercato. Recenti normative di recepimento di direttive comunitarie e delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas hanno obbligato l'ENI e le sue società controllate a programmare una progressiva diversificazione degli investimenti, volta a ridurre le sue quote nel mercato

congruenti con le proprie dimensioni aziendali. In dettaglio, il piano è articolato in più fasi. La prima fase, oggi in atto, prevede il trasferimento di titoli minerari a tre società, di recente costituzione, a capitale 100 per cento dell'ENI: Padana Energia, con sede a Marina di Ravenna, Adriatica Idrocarburi e Ionica Gas, con sede a Ortona. Le nuove società sono state costituite appositamente per ottimizzare lo sviluppo delle residue potenzialità connesse con i giacimenti conferiti, con particolare riferimento alla loro maggiore vicinanza al territorio, e sono state dotate di personale adeguato sia in termini di unità lavorative che di competenze tecniche. La cessione si configura come un «conferimento di ramo di azienda», costituito dalle quote di titolarità nei titoli minerari, unitamente al *know-how*, al personale e alle risorse tecniche e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività.

Nel periodo aprile-ottobre 2009, nell'ambito del processo di autorizzazione preventiva al trasferimento degli *asset*, l'ENI ha illustrato al Ministero tutte le fasi del processo, assicurando fin dall'inizio il mantenimento della piena occupazione dei lavoratori interessati. A seguito delle verifiche effettuate, attraverso l'esame dettagliato dei documenti presentati e delle integrazioni richieste, nell'ambito delle riunioni indette, è stato constatato che le società subentranti possiedono la necessaria capacità tecnica ed economica, così come prescritto dalla relativa normativa. Pertanto il Ministero dello sviluppo economico, in data 21 ottobre 2009, ha autorizzato preventivamente i richiesti trasferimenti, alle condizioni stabilite nella bozza dell'atto di cessione e nella convenzione in cui sono definiti gli impegni assunti da ENI in caso di inadempienza delle nuove società in caso di inadempienza delle nuove società agli obblighi di chiusura mineraria e ripristino dei siti. Si aggiunge, sulla base delle notizie fornite direttamente dall'ENI, che la stessa ha svolto una preselezione delle società interessate, per una eventuale cessione di due delle nuove società, Padana Energia e Adriatica Idrocarburi, ad altri operatori. Al riguardo, si sottolinea che anche per tali eventuali cessioni dovranno comunque essere espletate le prescritte procedure di autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, che vigilerà affinché sia garantito anche negli anzidetti eventuali trasferimenti il mantenimento della piena occupazione dei lavoratori coinvolti.

estremamente importante, perché porta chiarezza in un'operazione di strategia aziendale dell'ENI che potrebbe, per analogie con situazioni

abbiamo espresso delle critiche al riguardo - per come è stata condotta l'operazione Alitalia, con lo spacchettamento della *bad company* e della *new company*.

quindi ad incassare la polpa buona, scaricando la manodopera qualificata che vive ed opera all'interno di queste aziende. aziende. La risposta del Governo è importante. Resterà agli atti che il Governo, tramite le autorizzazioni che il Ministero dell'economia e gli altri Ministeri competenti concederanno,

sia i diritti dei lavoratori, in base ai contratti collettivi nazionali, sia gli stessi obiettivi aziendali e strategici di un settore così importante e delicato.

preliminare all'avvio del «Progetto di recapito», con la revisione globale del servizio. Tale fase di verifica ha interessato sia l'assetto dei servizi nelle varie Province, con l'individuazione e la delimitazione dei diversi bacini territoriali d'utenza, sia la definizione del dimensionamento dei centri corrispondenti a ciascun bacino. Nell'ambito del centro principale di distribuzione di Monza, l'organizzazione è stata completata e la copertura delle zone in cui sono ripartite le località accorpate, al momento, è assicurata dal personale di scorta e da unità assunte con contratto a tempo determinato. È stata riorganizzata la logistica interna e sono state individuate distinte aree di lavorazione, dedicate ad ogni singola attività. Ulteriori innovazioni sono state apportate anche alla sezione dedicata alla lavorazione della posta registrata: è stato infatti ottimizzato il *layout*, spostando la citata sezione nella nuova area del centro primario di distribuzione e curando la gestione dello sportello riservato alla corrispondenza inesitata. Inoltre, è stata individuata una specifica area di scambio del prodotto postale con un'agenzia partner per migliorare ulteriormente lo svolgimento del servizio di recapito. Nel centro secondario di distribuzione di Carate Brianza, grazie alle assunzioni a tempo indeterminato realizzate lo scorso 1° aprile ed alla definizione del *team* responsabile dell'ufficio, si sono sensibilmente ridimensionate le criticità verificatesi in passato, in buona parte riconducibili all'impiego di personale non di ruolo ed al frazionamento logistico-organizzativo dell'ufficio. I lavori alla struttura sono stati ultimati e i locali verranno consegnati entro la fine del mese di gennaio del 2010. A partire da tale data verranno individuate tutte le attività necessarie al trasferimento dei portalettere nel nuovo sito. Ai fine di consentire un maggiore presidio del territorio è al vaglio anche una modifica all'assetto, precedentemente previsto, dell'istituendo centro primario di distribuzione di Carate Brianza, che prevede l'accorpamento del presidio di Sovico al nuovo sito ed il mantenimento dei centro secondario di distribuzione di Giussano. È stato implementato poi il centro principale di distribuzione di Lissone, il centro di Biassono ha incluso i portalettere di Lesmo, Correzzana e Camparada, mentre il centro di Sovigo ha incluso gli addetti al servizio di recapito di Triuggio. Grazie a tali interventi le criticità evidenziate sono in via di progressiva risoluzione. Nel centro principale di distribuzione di Brugherio sono terminati i lavori di adeguamento previsti per i locali del centro primario di distribuzione e sono state concluse tutte le attività di accorpamento previste dalla nuova organizzazione: presidi decentrati di distribuzione di Agrate e spostamento dei portalettere di Concorrezzo dal centro primario di distribuzione di Vimercate al centro primario di Vimercate è stato reso operati e dotato del personale necessario. Peraltro, il Centro in parola, secondo Poste Italiane Spa, non presenta particolari problematiche, se non nei periodi di avvicendamento del personale a tempo determinato. Le lavorazioni interne registrano qualche disguido, in presenza solo di flussi di traffico di portata anomala, che comunque vengono prontamente fronteggiati, tramite il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

Sono stati incrementati vari settori grazie all'inserimento di 16 zone portalettere, all'applicazione di dieci unità di riferimento (un responsabile di Centro, tre *supervisors*, un addetto al monitoraggio e cinque capisquadra portalettere) e si è provveduto a 19 ulteriori stabilizzazioni di personale, nonché all'acquisto di 20 automezzi. Poste Italiane ha, inoltre, sottolineato che sono stati attuati, oltre a quelli già citati, interventi migliorativi di carattere immobiliare per il Centro principale di distribuzione di Meda, per le località di Monza, Desio, Limbiate, Carate Brianza, Giussano e Lissone. Inoltre, la sottoscrizione di una nuova locazione a Carate Brianza consentirà di riunificare l'omonimo Centro secondario con quello di Giussano. La nuova struttura assumerà l'organizzazione di un Centro principale di distribuzione con 43 zone portalettere e assicurerà il servizio di recapito nei comuni di Veduggio, Colzano, Renate, Briosco, Giussano, Verano Brianza, Besana presìdi saranno quindi portati da 14 a 9. La Concessionaria ha inoltre reso noto che, oltre alla rimodulazione degli orari di lavoro del personale, per ottimizzare lo svolgimento del servizio, tutte le zone dei Centri della Brianza sono state già dotate del nuovo casellario portalettere. Strumento che, oltre ad agevolare le attività preparatorie del servizio di recapito esterno, risulta particolarmente utile in caso di sostituzione del personale, fornendo, tra l'altro, informazioni relative all'elenco delle vie, dettagli attinenti al singolo civico, particolareggiate indicazioni di recapito riguardanti specifici clienti. La Concessionaria del servizio universale ha evidenziato, infine, che l'implementazione organizzativa del citato Progetto di recapito ha comportato un inevitabile quanto fisiologico periodo di difficoltà d'avviamento, ma che attualmente, nel contesto territoriale in esame, la situazione si presenta complessivamente in netto miglioramento. economico non mancherà comunque di verificare, tramite gli uffici competenti, che tale miglioramento sia reale e soprattutto che non si debbano più riscontrare i disagi riferiti dagli interroganti.

al problema in oggetto, mi permetto di evidenziare due aspetti sui quali, a mio avviso, il Ministero dovrebbe porre maggiore attenzione. I

da loro dovuti, a causa del ritardo dell'arrivo della posta. E non c'è ragione che regga. Le Poste hanno sbagliato e il cittadino - in questo caso, l'azienda - ha dovuto pagare o pagherà un'ammenda;

Ci sono invece casi in cui la consegna della posta in ritardo comporta danni di natura economica o disguidi che possono anche far incorrere in procedimenti penali.

sono elencati molti buoni principi (che in questa occasione mi hanno fatto sorridere): «Poste Italiane è presenza indispensabile per i cittadini, per le piccole e medie imprese, per le grandi aziende, per le amministrazioni pubbliche.

Grazie